L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'11 febbraio. Resta confermata per questa settimana la discussione del disegno di legge comunitaria 2010, a partire dall'odierna seduta pomeridiana. Nella seduta antimeridiana di domani, alle ore 12, saranno poste ai voti, a scrutinio segreto con procedimento elettronico, le dimissioni presentate dai senatori Cuffaro e Nicola Rossi. Le sedute della prossima settimana saranno dedicate all'esame del decreto-legge recante proroga di termini legislativi, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo si procederà alla calendarizzazione dei seguenti argomenti: disegno di legge sulla parità di accesso nei consigli di amministrazione delle società quotate, già approvato dalla Camera dei deputati; informativa del Ministro dell'interno sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari e sui flussi di ingresso; interrogazioni a risposta immediata - con la presenza del Ministro dell'ambiente - concernenti le ripercussioni sull'industria turistica dell'inquinamento nella zona di Napoli.

Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge comunitaria 2010 è stato presentato dal Governo il 5 agosto scorso, poco tempo dopo l'entrata in vigore della precedente legge comunitaria 2009, ed è stato assegnato alla Commissione politiche dell'Unione europea il 15 settembre. L'*iter* parlamentare di questo strumento legislativo si è quindi avviato avendo già in partenza accumulato ritardo rispetto a quanto prevede la legge n. 11 del 2005, cioè la legge Buttiglione, che disciplina le modalità della fase discendente, ovvero di attuazione degli obblighi che discendono dall'appartenenza all'Unione europea. Questo è dovuto al fatto di attendere la conclusione dell'*iter* relativo alla citata legge comunitaria del 2009. Strettamente legato al problema della dilatazione dei tempi è quello, lamentato da tutti durante l'esame della scorsa legge comunitaria, della progressiva ipertrofia dell'articolato del disegno di legge, che si è verificata in modo quasi sistematico Per avere contezza di ciò, basta vedere la differenza tra il numero degli articoli dell'iniziale disegno di legge rispetto al numero degli articoli con cui la legge è entrata in vigore. Parlo proprio del disegno di legge comunitaria del 2009, che era stato presentato in Parlamento con 9 articoli ma che è entrato in vigore con ben 55, diventando di fatto un vero e proprio *omnibus*. Durante l'esame invece di questo disegno di legge comunitaria, abbiamo cercato di porre un freno alle proposte emendative in base al criterio dell'oggetto proprio della legge comunitaria, così come definito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 e richiamato dal comma 4 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, ai fini della valutazione di ammissibilità dei relativi emendamenti, secondo il quale il contenuto della legge deve essere limitato a quelle norme direttamente connesse con la necessità di ottemperare a un obbligo attuale, ancora inevaso, derivante dall'ordinamento europeo. Certo, è spesso accaduto - e anche questa legge comunitaria non si sottrae - che il disegno di legge presentato dal Governo contenga *ab origine* delle disposizioni non direttamente o necessariamente rispondenti alla necessità di ottemperare a un obbligo attuale derivante o da atti comunitari non ancora recepiti o da procedure di infrazione ancora non risolte o da sentenze della Corte non eseguite. Ricordo però a tale riguardo che, mentre il comma 4 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento consente di effettuare un vaglio di ammissibilità per estraneità di materia sugli emendamenti, lo stesso non è previsto anche per il testo originario del disegno di legge, che quindi è giunto ad approvazione definitiva contenendo anche norme non rispondenti ai criteri che ho testé enunciato. per fare un esempio - si potrebbe dire che l'originario articolo 8 relativo alla nomenclatura europea di Roma capitale non non contiene una disposizione che risponde in maniera esplicita e diretta alla necessità di dare attuazione a un obbligo comunitario. Tuttavia, bisogna ricordare che una medesima proposta è stata fatta durante l'esame del disegno di legge comunitaria del 2009, per cui è comunque un argomento importante che è stato riproposto. Queste ed altre problematiche dovranno, per forza di cose, trovare un'adeguata sistemazione e una soluzione nell'ambito della riforma della legge n. 11 del 2005. Sappiamo che il Governo ha sue proposte e che sono stati presentati alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, sia alla Camera dei deputati, dove i testi sono in discussione, che al Senato della Repubblica. Peraltro, alcune modifiche della legge n. 11 del 2005 sono già state anticipate attraverso l'ultima legge comunitaria che ha introdotto gli articoli da 4-*bis* a 4-*quater* - concernenti l'attuazione degli atti di indirizzo delle Camere, il programma nazionale di riforma attuativo della strategia di Lisbona (ora strategia Europa 2020), la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e che ha sostituito l'articolo 15 contenente le relazioni annuali del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. A questo - permettetemi di ricordarlo - dovrà assolutamente essere aggiunta un'indifferibile riforma del Regolamento del Senato,

europea. Il 5 ottobre 2010 la Giunta per il Regolamento ha finalmente incardinato la trattazione di questo argomento: ci auguriamo pertanto che esso possa vedere al più presto la fine del

I, composto dagli articoli da 1 a 5, contiene disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,

al fine di assicurare un margine di tempo prima della scadenza del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva europea. Questo è dovuto alla prassi della Commissione europea,

che quasi in via automatica, già a distanza di un mese circa dalla scadenza del recepimento, viene inviata la lettera di messa in mora. Inoltre, è stato introdotto un nuovo comma 7, che attribuisce natura cedevole anche ai decreti legislativi recanti disposizioni sanzionatorie (evidentemente solo per le sanzioni amministrative) nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni.

la Relazione è già stata approvata dalla Commissione ed è agli atti. Mi limiterò pertanto a sottolineare due aspetti di ordine prevalentemente procedurale. Il primo riguarda la necessità e l'urgenza di provvedere

finestra"). Dichiaro aperta la discussione generale congiunta. La Presidenza informa che le proposte di risoluzione al documento LXXXVII, n. 3, potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

*(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, credo si imponga all'Aula una riflessione seria e chiara sullo strumento normativo sul quale noi oggi siamo chiamati a pronunciarci, se non vogliamo considerare la legge comunitaria annuale volta ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea come un semplice atto tecnico di *routine*. Una riflessione, quindi, credo si imponga, soprattutto di valenza politica, che deriva dalla necessità di cogliere anche questa occasione come momento per affrontare il dibattito sul ruolo dell'Italia nel processo di partecipazione all'Unione europea, su come concretamente e coerentemente lo realizziamo, su come il Parlamento si inserisce nel disegno di codecisione tracciato dal Trattato di Lisbona e sul ruolo che questo attribuisce al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Veniamo da mesi durante i quali, su questi temi, è stato importante il lavoro e il contributo svolto dalla 14a Commissione. Mi riferisco in particolare alla risoluzione sui rapporti tra Commissione europea e Parlamenti nazionali approvata lo scorso ottobre, al documento del Comitato presieduto dalla presidente Boldi istituito per adeguare il Regolamento del Senato alle nuove procedure europee, al piano nazionale di riforma attuativa di Europa 2020 all'indagine conoscitiva in corso sul sistema Paese con riferimento al ruolo del Parlamento nazionale nella formazione della legislazione comunitaria. Penso anche allo stesso lavoro prodotto nelle Sottocommissioni. C'è, insomma, un impegno e uno sforzo notevole, da parte della 14a Commissione tutta, cui il Gruppo del PD sta dando un contributo costruttivo, serio e prezioso, proprio per cercare di tessere il filo della consapevolezza della partita relativa al rafforzamento delle strutture comunitarie e per dare senso e valore alla nostra idea e al nostro modo di essere Europa e di costruire più Europa. Ma sono proprio queste considerazioni e quell'impegno che mi fanno dire oggi dell'urgenza di superare la debolezza e i limiti della legge comunitaria, già più volte e in diverse occasioni evidenziati. Limiti e debolezza che qui voglio, anche se in modo molto schematico, riprendere. La prima questione riguarda i tempi di approvazione della legge comunitaria. Il ritardo cronico è perfino imbarazzante:

Praticamente, stiamo sempre facendo un giro a vuoto. E così, mentre giovedì scorso si salutava con soddisfazione la riduzione del numero di procedure di infrazione aperte, il giorno dopo, il venerdì, giungeva la comunicazione di altre 24 procedure per mancato recepimento di direttive. L'altro aspetto è relativo all'esame congiunto di due strumenti così diversi fra loro quali la legge comunitaria e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, vanifica di fatto l'incisività. C'è poi la questione relativa alla crescente caratterizzazione della comunitaria come una delle tante leggi *omnibus* su cui attaccare di tutto ciò che ne depotenzia la funzione. Lo abbiamo visto lo scorso anno: da 9 a 55 articoli. Ha ragione la presidente Boldi: si è cercato questa volta di porre un freno, ma mi auguro che non si ripercorra la medesima esperienza dello scorso anno nei prossimi passaggi. Lo vediamo anche nelle materie trattate, alcune delle quali esulano dal contenuto proprio della legge comunitaria. Abbiamo sostenuto e sosteniamo, per esempio, come PD, la richiesta di stralcio dell'attuale articolo 12 (ex articolo 11), che introduce la delega al Governo per la disciplina della fiducia da inserire nell'ambito del codice civile. È assolutamente indispensabile e importante affrontare questa materia, anche per rispondere alle sfide della concorrenza fra ordinamenti. Ma rimane incomprensibile volerla introdurre attraverso la delega nella legge comunitaria, anziché intervenire con un disegno di legge specifico (e alcuni colleghi, del resto, ne hanno già presentati alcuni). Invito, oltretutto, tutti i colleghi, rispetto a questo articolo, a leggere il *dossier* del Servizio studi e la quantità di rilievi che esso pone su questa materia. Un'altra questione ancora è relativa all'ormai evidente inadeguatezza di questi strumenti, legge comunitaria e relazione, pensati e voluti per risolvere problemi in una fase emergenziale di recepimento della normativa europea e concepiti nel quadro dei precedenti Trattati. Strumenti, cioè, che per tempi, procedure, modi e ruolo del Parlamento sono stati calibrati utilizzando le lenti di lettura del passato e che ora necessitano di una rivisitazione complessiva. Il Trattato di Lisbona ha introdotto aspetti istituzionali di portata rilevante, relativi alle modalità di partecipazione dell'Italia al processo decisionale comunitario, in cui si privilegia, appunto, il momento del controllo parlamentare. Di fatto, però, gli strumenti che noi stiamo utilizzando ci consegnano, al contrario, una situazione rovesciata, con un evidente ruolo dominante del Governo e un depotenziamento dell'iniziativa legislativa del Parlamento in quanto tale. Presidente, colleghi, è a queste questioni che dobbiamo dare risposte urgenti: è sulla sempre più indifferibile esigenza di dotarsi degli strumenti giusti ed adeguati per poter agire con competenza, con maturità, con capacità, con qualità all'interno del processo democratico europeo che dobbiamo concentrare le nostre scelte. Non vediamo purtroppo - e lo dico con rammarico e preoccupazione - questa tensione positiva da parte del Governo. Non la vediamo in un Governo che pratica la completa dipendenza del Parlamento ai voleri dell'Esecutivo. Non la vediamo in un Governo che da mesi è senza Ministro per le politiche europee e di questo non se ne cura se non come opportunità per raccattare qualche eventuale voto. Non la vediamo in un Governo che spesso lancia messaggi contraddittori nel suo rapporto con l'Europa. E tutto ciò è tanto più drammatico in quanto ne va della credibilità del Paese, ne va della sua immagine, ne va della sua autorevolezza (già di per sé fortemente mortificate in questa fase). È per questi motivi che il Gruppo del Partito Democratico, con il senso di responsabilità costantemente dichiarato e praticato nei lavori di Commissione c'è e ci sarà convintamente nell'idea che gli adempimenti comunitari rappresentino l'asse portante di un modo di stare in Europa e nell'idea, soprattutto, di accettare l'Europa come fattore di cambiamento positivo per il nostro Paese. A Governo e maggioranza chiediamo chiarezza sulla volontà politica di perseguire questi obiettivi e chiediamo coerenza assumendo da subito le decisioni conseguenti.

l'oggetto della nostra discussione oggi, la legge comunitaria 2010, non fa eccezione al modello normativo che si è andato affermando in questa legislatura: una legge povera, in ritardo, poco innovativa e con disposizioni spesso estranee, purtroppo sempre estranee, all'oggetto proprio della legge. La legge comunitaria 2010 contiene cioè gli stessi vizi che hanno snaturato, nel 2008 e nel 2009, quanto quanto previsto dalla legge La Pergola, poi modificata dalla legge Buttiglione. È proprio questa incapacità, dimostrata dalla maggioranza e dal Governo, di correggere gli errori che porta il mio Gruppo ad avere una visione assai negativa di legge al nostro esame. Innanzitutto la tempistica della norma. È noto che il Governo dovrebbe presentare la legge comunitaria entro il 31 gennaio di ogni anno, in quanto la legge comunitaria è stata pensata come uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. È evidente tuttavia che tale periodico adeguamento non è sentito come una priorità dal nostro Paese, in quanto il Governo ha presentato il disegno di legge solo - lo sottolineo - il 5 agosto e lo stesso è stato assegnato alla 14ª Commissione permanente soltanto il 15 settembre. È evidente anche che questa maggioranza, che invece di porsi come interlocutore con il Governo agisce da suo braccio armato, non ha voluto accelerare il dibattito in Commissione in quanto la normativa arriva all'Aula ben cinque mesi dopo la presentazione, violando così quanto disposto dall'articolo 144-*bis* del nostro Regolamento che prescrive 30 giorni di termine massimo per il licenziamento dalla Commissione. Vorrei ricordare che siamo soltanto alla prima lettura, per cui, ad essere ottimisti, il disegno di legge verrà approvato alla Camera soltanto in primavera, cioè con un anno e mezzo di ritardo. Di tale inaccettabile ritardo, colleghi, è innegabilmente

Si tratta di un fatto gravissimo, che denunciamo fermamente, che ci pone fuori dalle prassi esistenti negli altri Paesi europei, nei quali nessun Governo si sognerebbe mai di lasciare il proprio Esecutivo senza il Ministro competente per le politiche comunitarie, soprattutto alla luce della sempre più crescente influenza di Bruxelles sull'economia, sull'ordinamento giuridico e sui diritti fondamentali, come il Trattato di Lisbona e la *governance* economica europea dimostrano. L'assenza di un Ministro responsabile politicamente davanti all'Europa e rispetto alla legge comunitaria, che oggi stiamo discutendo e che reca ancora la firma di Ronchi, è il segnale di quanta poca considerazione abbia Berlusconi per l'Europa.

su quanto poco valore il Premier dia al problema dell'Europa e delle risorse economiche che possono arrivare al nostro Paese, piegato dalla crisi (l'ISTAT oggi segna il punto più alto della disoccupazione giovanile: 29,9 se qui oramai tutto diventa un susseguirsi di ipotesi tragiche che, più si va avanti, più accelerano) e allo stimolo legislativo e politico a innovare, a crescere nei diritti e a proseguire sulla strada di una comunità di pace che ci viene dai Trattati, dalle direttive e dai regolamenti comunitari. Anche il contenuto della normativa riflette, dunque, la filosofia del Governo e il disprezzo che il Premier nutre verso l'Unione europea: non verso alcuni dittatori ma - ripeto - verso l'Unione europea. Il pericolo che avevamo ipotizzato, ossia che un disegno di legge molto snello fosse snaturato ed appesantito dall'approvazione di emendamenti tali da stravolgerne il contenuto normativo è stato confermato, è stato confermato, e durante l'esame in Commissione il provvedimento si è arricchito di ben 7 nuovi articoli, senza registrare praticamente quasi nessuna modificazione agli articoli contenuti nel testo originario. Questo è il risultato del fatto di aver approvato in Commissione ogni emendamento del Governo o del relatore che introduceva nuovi settori di regolamentazione, e di aver bocciato le proposte dell'opposizione, che invece volevano correggere in positivo il testo originario. Alla fine è uscito un provvedimento molto tecnico, che va a disciplinare, ad esempio, positivamente le concessioni per gli stabilimenti balneari, la professione della guida turistica o le tasse a carico dei produttori di dispositivi medici, ma che rimane restio ad affrontare i grandi temi. Mancano, infatti, temi fondamentali come l'immigrazione - in quanto ancora una volta è stata ignorata la direttiva che sanziona i datori di lavoro che si avvalgono di immigrati illegali - o come l'ambiente. E non possiamo stupirci, visto che la relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea, alla sezione III (energia e cambiamenti climatici), dà conto di come il Governo abbia dimostrato poco coraggio nel perseguire gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni inquinanti, mancando di individuare incentivi per le industrie con compatibilità ecologica, e come abbia rappresentato anzi un freno per gli Stati membri più avanzati in materia di implementazione della politica ambientale e nel raggiungimento del cosiddetto accordo 20-20-20, per il quale ha anche avanzato una proposta di riforma che ne riduce l'apporto. A fronte di questi vuoti rilevanti, si annoverano invece dei provvedimenti che fungono da *spot* per il Governo: il regalo ad Alemanno con l'articolo 8 su Roma capitale, che crea uno *status* della capitale senza nessuna determinazione dei poteri e delle funzioni del nuovo organismo, rischiando di renderci ridicoli presso l'Unione europea, in quanto sarebbe stato giusto affrontare seriamente cosa fa Roma capitale e come lo fa, prima di chiedere a Bruxelles di aumentare i finanziamenti con la rideterminazione del livello NUTS il regalo a Finmeccanica, all'articolo 16, dove, ignorando il dibattito che si svolgeva presso le Commissione affari esteri e difesa, nel recepire la direttiva sul commercio e il transito di armi, si prevedono sanzioni per reati connessi al traffico di armi di carattere penale o amministrativo con una multa che al massimo arriva a 150.000 euro, rischiando così una depenalizzazione gravissima di tali reati, con conseguenze catastrofiche in termini di sicurezza e lotta alla criminalità organizzata. Su questo c'è stato silenzio. Insomma, dalla legge comunitaria non escono nuovi diritti e non vengono affermate nuove frontiere sull'uguaglianza, ma il Governo ha scelto con certosino calcolo le disposizioni che evitano qualsiasi scontro politico e ha privato dei risvolti più profondi e più europei le direttive in analisi. Penso, ad esempio, all'articolo 10 della legge comunitaria, ove, nel recepire le direttive sulle telecomunicazioni e sulle comunicazioni elettroniche, è stato fatto calare ad arte il silenzio sul distorto sistema italiano. Non vorrà dirmi infatti il Governo che nel nostro sistema oligopolista, con la tv pubblica in mano ai politici, con le tv private proprietà del *premier* e con i concorrenti come Sky balzellati ad arte per renderli meno competitivi, esiste quella parità di accesso al mercato con i criteri di obiettività e non discriminazione che invece sbandiera al comma 3 della lettera *a)*! O vorrà forse sostenere che siano stati attuati che siano stati attuati gli strumenti per garantire che i disabili sensoriali abbiano accesso all'informazione, come invece proclamato al comma 3 della lettera *f)*, quando alla RAI ancora non è stato bandito il concorso per offrire il servizio di sottotitolazione, mentre negli altri Paesi europei ogni programma di informazione, telegiornale o approfondimento viene sottotitolato? Ecco perché, se questa deve essere una legge comunitaria obsoleta e poco ambiziosa, allora non posso non concordare con le proposte avanzate dai colleghi dell'opposizione (dalla senatrice Marinaro in particolare, che ringrazio per la sua esperienza e per i suoi suggerimenti, e qualche volta per le bacchettate che mi dà) riguardo alle riforme sui meccanismi di adeguamento del nostro sistema normativo a quello europeo. Dobbiamo pensare a provvedimenti *self executing* per le direttive cosiddette tecniche, che poco abbisognano della riflessione del Parlamento e che soprattutto non possono attendere un anno e mezzo prima di essere recepite, rischiando di incorrere in costose procedure di infrazione, e dobbiamo concentrare la nostra attenzione su quelle di maggior rilievo politico e giuridico, che in questa legge comunitaria mancano totalmente. Mi avvio alla conclusione chiedendo che il Governo prenda atto di queste parole e responsabilmente accolga i suggerimenti che dall'opposizione arrivano tramite gli emendamenti e gli ordini del giorno che ci apprestiamo a discutere, non solo sul contenuto del testo ma anche sulle procedure. Soprattutto, il Governo non sottovaluti la responsabilità politica di lasciare

respiro, troviamo adempimenti che riguardano politiche sociali ed immigrazione, questioni finanziarie, fino all'applicazione di regole nel settore delle comunicazioni. È su queste ultime che intendo soffermarmi brevemente per svolgere qualche considerazione. L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepire le direttive del Parlamento europeo relative al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione. vi si legge, tra l'altro, che il Governo sarà impegnato a garantire accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Si parla di gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza e in linea con i princìpi di neutralità tecnologica dei servizi. Si parla poi di rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e si prevede poi l'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica. Potrei andare avanti a lungo, perché questo articolo 10 è corposo e pieno di promesse interessanti: tuttavia, è lecito domandarsi se stiamo scrivendo una legge o un semplice elenco di buoni propositi, visto l'atteggiamento dilatorio, se non addirittura omissivo, che il Governo ha fino ad ora tenuto in questo delicato settore. Il problema non è la qualità della delega, ma la qualità del delegato. Basta pensare allo strano fenomeno carsico che ha riguardato i famosi 800 milioni di euro destinati alla banda larga, comparsi e poi scomparsi nelle diverse leggi finanziarie, finanziati e definanziati a seconda di come tirava il vento e, in buona sostanza, passati in cavalleria o fortemente a rischio di passare in cavalleria, visto che oggi,

del CIPE. A parole sosteniamo di condividere gli impegni europei, quel piano che prevede la copertura totale della banda larga cosiddetta *light* in tutta la popolazione nel 2020; però, obblighiamo i medici di base a inviare i certificati per via elettronica - basta leggere «Il Sole 24 Ore» di oggi sull'argomento - salvo scoprire che i poveretti non sono in grado di ottemperare a questo obbligo, non già perché privi di *computer* ma perché privi in gran parte del Paese delle infrastrutture di trasmissione adatte. Intanto, il Ministero dell'economia guarda con grande interesse all'asta delle frequenze liberatesi con l'introduzione del digitale terrestre, non già per reinvestirne gli introiti per finanziare la crescita del settore della comunicazione, ma solo per acquisirli e riversarli a parziale sollievo del debito pubblico. Sono solo piccoli e marginali episodi questi, o sono l'ennesima prova del fatto che stiamo trattando l'Europa, le sue istituzioni, le sue regole come in casa si tratta il vecchio zio saggio, che però è noioso e a cui si dà ragione per evitare di sostenere barbose discussioni? Davvero questo Governo sarà così sollecito e zelante da seguire le indicazioni dell'Europa su un settore che, tra l'altro ‑ lo dico a bassa voce ‑ sta particolarmente a cuore al Presidente del Consiglio e alla di lui famiglia? È lecito dubitare. Ma è lecito coltivare dubbi a tutto tondo sul vero sentimento europeista di questo Governo: lo ha già detto chi mi ha preceduto. Senza nulla togliere all'autorevole Sottosegretario che siede ora sul banco del Governo, è il caso di ricordare che dopo le dimissioni del ministro Ronchi non si è evidentemente avvertita la necessità né l'urgenza di sostituirlo. sostituirlo. In Commissione 14a, per esempio, abbiamo avuto il piacere negli ultimi mesi di interloquire, ora con un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ora con un Sottosegretario agli esteri: tanto, la delega si può trasferire. Mi domando se anche nelle riunioni di Bruxelles e Strasburgo siamo rappresentati allo stesso modo. Chiudo così il mio intervento: le domande restano sicuramente senza risposta, come al solito, e così restano le nostre perplessità sulla vera utilità e sulla reale applicabilità di quanto previsto da questo provvedimento.

al rinnovo automatico delle concessioni, alla modifica del Testo unico finanziario, e poi alla questione che riguarda gli organi di investimento collettivo di valori mobiliari. Ci sono alcuni articoli che, in effetti, sono stati introdotti. Alcuni di essi ‑ ne ha parlato anche chi mi ha preceduto, in particolare il senatore Pedica ‑ riguardano la sanatoria. In ogni atto c'è una sanatoria che il Governo deve fare. Anche il

l'articolo 7, al fine di armonizzare la legislazione nazionale al dettato comunitario, apporta modifiche - a quattro articoli del codice del consumo in materia di servizi finanziari. La prima modifica riguarda l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro La seconda modifica interviene sul diritto di recesso, espungendo dal testo oggi in vigore l'inapplicabilità di detto recesso ai contratti di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore.

per penalizzare ancora una volta i consumatori che sono stati già ampiamente vessati dalle compagnie, che applicano in Italia tariffe più alte d'Europa nel settore della RC Auto,

Sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, è opportuno ricordare che, nell'ordinamento interno, il quadro di riferimento in materia è la disciplina dettata dal Testo unico delle

in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate, hanno la finalità di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta al rispetto delle norme italiane sulla costituzione ed il funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, mentre la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio in Italia da parte di succursali delle società di gestione armonizzate rispetti le regole di comportamento

la procedura di infrazione 2008/4908 ai danni dell'Italia, la Commissione europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni sul demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative

è stato sollecitato a venire in quest'Aula per proporci gli ultimi rantoli di un regime ormai pronto a passare a miglior vita. In quell'occasione, con il pretesto di parlare di politica estera, il ministro Frattini si è prestato ad una delle tante vergognose azioni di depistaggio o di costruzione di scenari inquietanti, venendo qui a parlare di Santa Lucia piuttosto che di ciò che sta accadendo nel nostro Paese. E dunque, la trattazione di questo argomento, colleghi, avviene in un momento particolare, sia per l'Italia che per il resto del mondo. Nel resto del mondo - mi riferisco in particolare al Nord Africa - stiamo assistendo ad una straordinaria mobilitazione per la democrazia di quei Paesi; e se da una parte vediamo una intelligente e lungimirante apertura degli Stati Uniti d'America nei confronti di quei Paesi (apertura che si è determinata nonostante rapporti solidi di amicizia che quello stesso Paese nordamericano ha stabilito per decenni con gli altri del Nord Africa) non c'è stato alcun tentennamento di fronte a questo anelito di democrazia. L'Europa, invece, ritarda, tentenna, indugia e, tanto per cambiare, se l'Europa tentenna e indugia in Italia non se ne parla neppure. In Italia ci sono altre cose di cui occuparsi: le questioni

ci vuole molta bonomia per fare in modo che il dibattito odierno si possa sviluppare anche con una visione di merito rispetto alle cose, senza farsi condizionare troppo - benché sarebbe assolutamente comprensibile - dal clima da fine impero che sta ammorbando il nostro Paese. Vorrei fare, inoltre, alcune considerazioni più specifiche rispetto alla materia della quale comunemente mi occupo. Vorrei parlare dei problemi della difesa. Cari colleghi, a voi è noto che, il pretesto di trasformare questo provvedimento legislativo in un provvedimento *omnibus*, in una sorta di calderone in grado di poter ospitare tutto e il contrario di tutto, come altri colleghi hanno già già avuto modo di dire, si è tentato il colpaccio. E devo dire che si deve anche alla cortesia istituzionale della Presidente della Commissione e allo stesso sottosegretario Scotti qui presente se

che si intendeva realizzare. Gabellando il provvedimento per qualcosa che potesse in qualche modo rientrare nella legge comunitaria, si voleva immettere, con una norma vergognosamente intrusa, tutto un armamentario - è proprio il caso di dirlo - di tipo pseudolegislativo per permettere di commercializzare le armi senza un minimo controllo da parte del Parlamento. ciò è stato evitato: questo tentativo è stato sventato. Però c'è stato. Il vizio di utilizzare il Parlamento soltanto per obiettivi funzionali a determinate esigenze e a determinate prospettive, come vedete, non viene mai meno. Sempre per restare in materia, va detto che, nonostante il Trattato di Lisbona, nonostante questa importantissima novità in termini di governo sovranazionale, piuttosto che alla cooperazione strutturata permanente, che il medesimo trattato suggerisce, il presidente della Repubblica Napolitano ci ha non più tardi del luglio 2010 - leggo testualmente - «ad alleggerire i bilanci nazionali dei Paesi membri, eliminando le duplicazioni di spesa oggi esistenti». Tutto questo, però, signora Presidente, colleghi, non è piaciuto al nostro Governo di turno,

lo spirito della legge comunitaria vada ripreso e rilanciato e, per quanto attiene nello specifico alle questioni legate alla difesa e alla sicurezza siamo del parere, già espresso in una mozione approvata all'unanimità, che si debba procedere con decisione verso la costruzione di uno strumento militare comune europeo, nel segno della riduzione degli armamenti e dell'implementazione di tutte le risorse finalizzate alla cooperazione e allo sviluppo. Allora parlare d'Europa non sarà soltanto una finzione, ma sarà il sostanziare concreto di un'ispirazione che parte da molto lontano. la discussione della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 cade in una fase storica molto particolare. Nel 2009 la crisi economica ha continuato a far sentire i propri effetti. Dopo il crollo del prodotto interno lordo registrato nel 2008, lo scorso anno abbiamo assistito ad una sostanziale stagnazione in quasi tutti i Paesi, Italia inclusa, che ha provocato un drastico aumento del numero dei disoccupati. C'è stato un peggioramento della disoccupazione minore rispetto a quella riscontrata negli Stati Uniti, investiti in pieno dalla crisi, ma comunque ragguardevole, visto che il tasso di disoccupazione in Europa è passato da poco più del 7 per cento degli anni 2007-2008 a oltre il 9 per cento nel 2009. Anche le finanze pubbliche in Europa hanno subito un notevole deterioramento. L'indebitamento netto nella media dei Paesi

la moneta unica si è trovata a fronteggiare una situazione di potenziale *default* di uno Stato sovrano appartenente all'area valutaria. Sarà ricordato come l'anno della crisi del debito greco e solo di quello greco, per fortuna. La crisi internazionale in atto si accompagna ad un quadro geopolitico mondiale che rimane tuttora molto complesso ed estremamente fluido, cosa che impone alle istituzioni comunitarie e a tutti i Paesi membri una profonda riflessione sul ruolo dell'Unione europea nel contesto mondiale, riflessione che deve essere produttiva però di effetti concreti, soprattutto in tema di affari esteri e di politica della sicurezza. Questa situazione ha imposto il varo di importanti provvedimenti a livello comunitario. Si è trattato di provvedimenti in materia di regolamentazione dei mercati finanziari, di misure di urgenza per fronteggiare eventuali nuove crisi dei debiti sovrani nei Paesi dell'area dell'euro. Alcuni di questi interventi, anche a causa di concomitanti scadenze elettorali in qualche Paese membro, sono giunti in porto dopo un *iter* molto travagliato. Basta ricordare la creazione del fondo salva-Stati. In secondo luogo, l'Europa ha provveduto ad una importante riforma dei trattati istitutivi, riforma che ha tenuto conto in modo notevole del nuovo quadro interno ed internazionale emergente dalla crisi. Il nuovo Trattato di Lisbona, entrato in vigore il primo dicembre 2009, ha innovato profondamente l'organizzazione, le competenze e le strategie della UE. Per quanto riguarda gli aspetti dell'emergenza economica e finanziaria, molto lavoro è stato svolto dall'Ecofin in tema di coordinamento delle politiche economiche contro la crisi, con il chiaro obiettivo di rilanciare la crescita e aumentare l'occupazione. Sempre in sede di Consiglio Ecofin sono state poi approvate le linee generali per l'istituzione delle tre ESA (*European* *Superivisory* *Authority*), ovvero le tre nuove importanti autorità di vigilanza sui servizi e sui mercati finanziari in ambito UE. Sono state avviate molte procedure per disavanzi eccessivi. E anche l'Italia è stata destinataria di raccomandazioni circa il rientro del disavanzo pubblico sotto il 3 per cento entro il 2012.

Una riforma che integra e rafforza lo storico Patto di stabilità e crescita. In particolare, poco si è detto sulla reale portata di tale riforma e sulle conseguenze in termini di discrezionalità e spazi di manovra per le politiche economiche dei singoli Paesi membri. Poco si è detto circa le conseguenze per la politica di bilancio in un Paese come l'Italia, sia sul processo di programmazione con l'introduzione del semestre europeo, sia sui contenuti dei provvedimenti. Per quanto riguarda i nodi strutturali dell'economia, gli impegni dell'Unione europea si sono concentrati da un lato sul tema del costo e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e dall'altro sul miglioramento del mercato interno. Per quanto riguarda in particolare il tema del mercato interno dell'energia, l'istituzione dell'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è un passo importante verso la creazione di una unica rete europea dell'energia. In questo senso il nuovo regolamento europeo in tema di infrastrutture energetiche definisce principi sulle tariffe, sui servizi offerti, sull'assegnazione della capacità, la trasparenza e il bilanciamento delle reti. Lo sviluppo della *green economy* è uno degli obiettivi più rilevanti e innovativi inclusi nella strategia «Europa 2020». Anche qui, nel merito della relazione, va sottolineato che con un po' più di coraggio si sarebbero potuti individuare obiettivi prioritari più precisi per gli anni a venire, sia per quanto riguarda lo sviluppo della *green economy* e delle energie rinnovabili, sia per quanto riguarda le fonti tradizionali. Il 2009 è stato anche l'anno della conferenza di Copenhagen sul clima. Su questo tema dobbiamo rilevare che purtroppo proprio il vertice di Copenhagen, che avrebbe dovuto sancire il ruolo di *leader* mondiale dell'Unione europea sul tema delle politiche contro i cambiamenti climatici, si è rivelato molto al di sotto delle aspettative. E questo nonostante il corposo impegno normativo dell'Unione europea e dei Paesi membri. In questo senso, anche le ambizioni del Governo italiano hanno seguito a ruota il destino di quelle europee.

Proprio sul tema dell'impegno italiano alla riduzione delle emissioni di C02 è il caso di richiamare l'attenzione sulla necessità di pervenire a un nuovo accordo, con un impegno più equilibrato per il nostro Paese, che tenga conto di una effettiva analisi costi-benefici delle politiche assunte. Anche perché Paesi grandi come gli USA e la Cina in tema di riduzione delle proprie emissioni hanno autonomamente assunto impegni molto meno vincolanti, se rapportati alla dimensione assoluta delle loro economie. Va aggiunto poi che le reali risultanze scientifiche sul tema delle emissioni di C02, sulle loro cause, sulle loro conseguenze e soprattutto sul reale impatto delle politiche di riduzione sul cambiamento climatico non sono affatto chiare e univoche. A tale proposito troviamo quanto mai opportuno che l'Italia si faccia promotrice nelle sedi internazionali di iniziative di studio e ricerca, mirate ad approfondire gli aspetti scientifici del cambiamento climatico, contribuendo a fare chiarezza su un tema così complesso e sul quale negli ultimi decenni si è fatta anche molta speculazione ideologica. Molto importante, sotto il profilo della politica estera comune europea, è stata la revisione della figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al quale vengono affidate una serie di funzioni che prima afferivano separatamente al Commissario per le relazioni estere e all'Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune. L'Alto rappresentante diventa anche vicepresidente della Commissione europea. Secondo i dati riportati nella relazione è migliorata la *performance* del nostro Paese nel recepimento delle normative europee. Il *deficit* dell'Italia nel recepimento delle direttive comunitarie, pur restando ancora distante dall'obiettivo dell'1 per cento fissato nel 2007, si è ridotto passando dall'1,7 per Anche per quanto riguarda le procedure di infrazione, pare che a fine 2009 si sia registrato il più basso tasso di procedure pendenti; ma anche a tal riguardo siamo distanti dagli *standard* dei nostri *partner* europei. Pertanto, lo sforzo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea non può certo fermarsi, ma deve continuare. Quest'ultimo tema acquista ancora più importanza in fase di approvazione della legge comunitaria 2010. Anche noi riteniamo ormai indifferibile una modifica al Regolamento del Senato, quale attribuisca alla 14a Commissione prerogative e funzioni adeguate al compito non solo di recepire le leggi europee nell'ordinamento italiano, ma anche di monitorarne l'effettiva implementazione ed il coordinamento sistematico tra la normativa nazionale e quella comunitaria. L'ordinamento nazionale sempre più di frequente deve essere adeguato a normative europee che sono numerose, complesse e soprattutto pervasive, tanto nei diversi settori dell'economia quanto ormai nella vita dei cittadini. Vogliamo anche esprimere l'auspicio che la legge comunitaria divenga finalmente lo strumento attraverso il quale il Governo entri nel merito delle questioni investite dalla normativa comunitaria, e non sia una semplice lista di adempimenti formali. Questo, ovviamente, richiede competenza, coerenza, coraggio e volontà politica di scegliere.

e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è un passaggio importante dell'attività legislativa, perché consente, da un lato, di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario di verificare il coinvolgimento nazionale nella costruzione europea. Per quanto attiene alla legge comunitaria, non ripeto le puntuali osservazioni espresse dai colleghi senatori che mi hanno preceduto in merito al grande ritardo dell'esame del provvedimento. Non può questo fatto non essere qualificato come scarsa attenzione del Governo e della maggioranza alle esigenze dell'Unione europea. Sottolineo invece che il Partito Democratico ha sempre tenuto un comportamento di alta responsabilità nei confronti della legge in argomento. Ha espresso concordanza e condivisione allorché le proposte evidenziavano la corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale degli indirizzi politici dell'Unione europea. Ma ha anche denunciato con forza le interpretazioni della legge difformi dallo spirito del Trattato di Lisbona, come quando sono state inserite norme non in armonia, se non addirittura in contrasto, con i principi comunitari, oppure quando si è cercato di proporre nel provvedimento tematiche che nessuna attinenza avevano con la legge comunitaria. Nell'analogo provvedimento dello scorso anno, per esempio, la visione del Governo di non recepire norme europee relative al fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare, e di emendare la legge comunitaria con temi che richiedevano invece uno specifico coinvolgimento da parte del Parlamento, ha costretto il Partito Democratico a votare per la prima volta contro la stessa legge comunitaria. Sicuramente, anche per questa azione risoluta, la legge comunitaria relativa al 2010, quella che oggi esaminiamo, presenta aspetti meno censurabili. Innanzitutto il disegno di legge contiene essenzialmente provvedimenti inerenti alla materia comunitaria. Il Governo ha evitato in sostanza di ricadere nella tendenza a trasformare la legge comunitaria in un provvedimento *omnibus*, ossia in uno strumento per inserire nell'ordinamento nazionale norme completamente estranee alla materia in esame. Inoltre, soprattutto grazie all'azione del Partito Democratico, si è evitato di ampliare strumentalmente le deleghe al Governo in tematiche che necessitano invece di un attento esame del Parlamento. È testimonianza di ciò il mantenimento dell'integrità della legge sull'esportazione e il transito dei materiali di armamento, la quale non poteva essere modificata, come inizialmente tentato dal Governo, nel momento di recepire una norma relativa ad un aspetto molto circoscritto del settore. In conclusione, la legge comunitaria per il 2010, che è il provvedimento più importante della discussione odierna, presenta una evoluzione positiva rispetto a quella relativa all'anno precedente e il Partito Democratico è stato senz'altro promotore con le sue sollecitazioni e i suoi richiami nell'ottenere questo importante risultato. Non posso peraltro non sottolineare il fatto che il provvedimento, nel prosieguo del suo *iter* legislativo, potrebbe incorrere nelle gravi distorsioni di cui ho parlato. Il giudizio definitivo potrà essere dato quindi solo al termine di questo cammino; ma sarebbe molto grave se il Governo, per ragioni politiche di parte, dovesse di nuovo inquinare ingiustificatamente e pericolosamente una legge finalizzata alla costruzione dell'Unione europea.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la legge comunitaria, così come viene proposta e così com'è impostata, ancora una volta non può che essere considerata un atto burocratico, un atto tecnico. Ancora una volta, essa viene presentata con oltre un anno di ritardo; ancora una volta, essa presenta un'impostazione che mette insieme direttiva per direttiva; ogni singola misura è presa a sé, al di fuori di un contesto e slegata da una politica. che questo non ci aiuti a capire quali sono non tanto le direttive, quanto piuttosto le direzioni verso cui l'Unione europea intende andare sulle grandi questioni del lavoro, dell'ambiente, delle comunicazioni, del commercio, delle migrazioni dei cittadini e delle loro nuove integrazioni,

tratta di uno scarto insopportabile, che rende vana questa nostra discussione. Nel settore agricolo, forse più che in altri, si avverte questa distanza. L'agricoltura è quel settore che ha costituito l'elemento fondante dell'Unione europea; gli imprenditori agricoli sono stati i primi cittadini europei. l'agricoltura è questione centrale; oggi dire agricoltura significa dire cibo, salute, ambiente, energia, cultura, lavoro con alti costi oppure, al contrario, lavoro nero con sfruttamento fino allo schiavismo. L'agricoltura di una complessità che stiamo vivendo in questo tempo, in questa nostra Europa. Non cogliere l'occasione della legge comunitaria, modificarne l'impostazione e l'importanza per un confronto sulle scelte e sugli obiettivi, è visione miope; è l'atteggiamento di chi subisce l'Europa e non di chi crede in un bisogno di più Europa oggi. Sì, la legge comunitaria è strumento per il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario; così sta scritto. Ma questo non significa che si tratta di un automatismo tecnico e che non si deve cogliere l'occasione degli adeguamenti per risalire alle scelte politiche, alla cornice che li accoglie e che permette ai Parlamenti di intervenire davvero sulle politiche. Per questo è nato il Trattato di Lisbona, per dare un impulso notevole al ruolo dei Parlamenti nazionali. E, se proprio l'articolo 12 del Trattato sancisce che «i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione», credo che questa modalità, che si protrae stancamente nella discussione della legge comunitaria, non corrisponda a questo fine. Non mi soffermo sui singoli punti che riguardano specificamente la materia agricola e il settore alimentare e ambientale, come le direttive sui succhi di frutta, le sementi foraggere, l'uso sostenibile dei pesticidi, l'importazione da Paesi terzi di pollame e uova, queste ultime al centro di preoccupanti fenomeni di contraffazione. Non è questo il luogo e non c'è tempo per entrare nel merito. Sui singoli punti il Gruppo PD in 14a Commissione ha contribuito in modo importante e, in alcuni casi, è stato decisivo perché non si allargassero le maglie relative alle garanzie e al rispetto della sicurezza alimentare. Così come abbiamo convenuto sull'articolo 18, perché siamo tra coloro che vogliono incentivare e promuovere un processo di modernizzazione nel settore della pesca, pur consapevoli delle gravi difficoltà che questa questa riconversione comporta proprio per l'adeguamento alle normative europee. Proprio per questo, ci siamo fatti promotori di un emendamento e di una richiesta di incremento delle risorse destinate al settore nell'ambito del provvedimento milleproroghe, che andremo a discutere tra qualche giorno. Abbiamo lavorato perché in ogni direttiva venisse sancito in ogni direttiva venisse sancito il diritto dei consumatori a conoscere e ad essere messi in condizione di poter verificare la tracciabilità del prodotto. Si tratta della stessa convinzione che ci ha portato a condividere la legge sull'etichettatura, che, ancor prima di una vertenza sulle norme in Europa, è un confronto culturale di alto senso civico e di diritto alla conoscenza di cui questo Paese vuole farsi interprete. Vorrebbe essere traino di processi normativi che diano ai consumatori europei nuove libertà di scelta e nuovi poteri di condizionare i mercati verso parametri di alta qualità negli alimenti. Per questo, non si può discutere di una somma di direttive come se fossero sospese nel vuoto. Non si può ignorare che, mentre registriamo alcuni adeguamenti normativi, parallelamente e contemporaneamente, in Europa, si sono conclusi provvedimenti che ne modificano la portata. Mentre ragioniamo di un singolo prodotto e della sua presente collocazione sul mercato, si sta concludendo il pacchetto qualità che racchiude modalità, impostazioni e indirizzi sulle produzioni alimentari, sui prodotti tipici, su parametri della loro composizione: provvedimenti sulla ricerca, sulle politiche di coesione, sulle politiche commerciali, con conseguenze dirette su alcune filiere produttive europee. Senza dimenticare che da un anno ormai a Bruxelles, come in ogni Paese membro, si sta discutendo delle nuove linee della Politica agricola comune, la PAC, che mette in discussione una visione che collega alimenti, salute, salubrità ambientale, salubrità ed etica del lavoro. Mi chiedo se noi possiamo permetterci di fare una disamina utile e concreta sulla legge comunitaria, con una discussione che esula e si estranea da tutto questo. Chiediamoci se tutto questo ha un senso e se crediamo davvero nel futuro dell'Europa.

che lo rende particolarmente interessante. Potrebbe infatti essere l'ultimo, o uno degli ultimi, approvati secondo il modello di legge comunitaria ideato sin dalla cosiddetta legge La Pergola del 1989, cioè secondo il modello della delega legislativa al Governo. Lo strumento della legge comunitaria è stato oggetto di una particolare attenzione in questi ultimi anni da parte degli operatori, del Governo e del Parlamento, perché è divenuto lo strumento principale attraverso il quale rendere funzionale l'attività delle istituzioni parlamentari e governative al tempestivo recepimento della normativa europea. Attraverso la legge comunitaria annuale si è cercato di dare una concretezza maggiore al rapporto fra l'ordinamento interno e quello sovranazionale europeo, che ha vissuto momenti di tumultuosa evoluzione in questi anni e che ha trovato difficoltà nella fase di recepimento. Tuttavia, non sempre la legge comunitaria si è dimostrata adeguata allo scopo cui è destinata. Infatti, in alcuni casi particolarmente rilevanti è stato necessario adottare strumenti d'urgenza, tali da sopperire ai talvolta lunghi *iter* caratterizzanti l'esame parlamentare della legge comunitaria. Mi riferisco ai cosiddetti decreti anti-infrazioni, emanati a più riprese per consentire il veloce adeguamento alla normativa comunitaria, reso indifferibile dalla possibilità concreta di essere chiamati a risponderne innanzi alla Corte di giustizia, sotto comminatoria di consistenti ammende comunitarie. Questi strumenti si sono resi necessari per dare risposta a una duplice esigenza: quella di una risposta al mercato, che chiede alle istituzioni nazionali un pronto recepimento delle norme comunitarie e, dall'altra, quella di una risposta alle istituzioni comunitarie che ci impongono un adeguamento corretto e nei termini, al fine di permettere quell'integrazione tra ordinamenti che è la base stessa della Costituzione europea. Per far fronte al problema del recepimento in modo strutturato, occorre quindi voltare pagina, non solo rispetto alla comunitaria come l'abbiamo conosciuta, ma anche rispetto alla produzione normativa per decreto-legge. Tenendo conto di questo quadro di riferimento, il 16 novembre 2010, il Governo, con il suo ora ex ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, ha presentato un organico progetto di legge di riforma della cosiddetta legge Buttiglione, che attualmente è in discussione alla Camera e in cui è contenuta una importante novità per quanto concerne i provvedimenti di recepimento della normativa dell'Unione europea. L'articolo 19 del progetto di legge, infatti, prevede due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea. Si tratta, in sostanza, di uno sdoppiamento del disegno di legge comunitaria, in un primo disegno di legge da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, che reca esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all'autorizzazione in via regolamentare, e un secondo disegno di legge da presentare al Parlamento, anche disgiuntamente rispetto al primo, che reca disposizioni di attuazione diretta. Come ha rilevato lo stesso ministro Ronchi nell'audizione svolta al Senato il 19 maggio 2010 sull'attuazione del Trattato di Lisbona, appare indispensabile velocizzare gli strumenti attualmente in uso per arrivare al recepimento della normativa europea. europea. Infatti, la legge comunitaria sta mostrando dei limiti sotto questo profilo, considerando la sua crescente caratterizzazione come legge *omnibus*, che costringe il provvedimento a ripetute *navette* tra i due rami del Parlamento. Non è questa la sede per valutare l'impostazione offerta dal progetto di legge governativo: il problema della lunghezza dell'*iter* procedurale della legge comunitaria, comunque, è stato più volte sollevato nel corso dei lavori parlamentari. Possiamo dire però che la legge comunitaria è stata ed è uno strumento utile che ha fatto la storia della legislazione in Italia. Ora occorre però un nuovo approccio. Per quanto riguarda il testo, vorrei soffermarmi sull'articolo 8, che riguarda la materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. La direttiva adottata nel 1985 mirava ad offrire maggiori opportunità, sia agli operatori del settore sia agli investitori, integrando il mercato dell'Unione europea dei fondi di investimento. È stata fondamentale per lo sviluppo dei fondi di investimento europei ed ha subito diverse e sostanziali modifiche. In occasione delle ultime modifiche, che tendono ad adeguare il quadro giuridico degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai mercati finanziari del 21° secolo, per ragioni di chiarezza, si è proceduto alla sua rifusione. Nell'ordinamento interno il quadro di riferimento è la disciplina dei fondi comuni di investimento, cosiddetti armonizzati. Le modifiche normative proposte sono necessarie per assicurare il pieno funzionamento del cosiddetto passaporto delle società di gestione, che ora permette a queste ultime di costituire fondi comuni in un Paese membro dell'Unione europea diverso da quello di origine e, oltre a ridefinire l'operatività transfrontaliera, vengono attribuite a CONSOB e Banca d'Italia poteri di vigilanza e di indagine.

al risparmio gestito, che tassa i risultati maturati. Questo è un vecchio problema che ci siamo posti varie volte: ho anche presentato un disegno di legge per arrivare ad una armonizzazione tra la nostra normativa e quella degli altri Paesi europei, quindi per passare dalla tassazione sul maturato alla tassazione sul realizzato. Un altro punto importante riguarda l'articolo 11. A questo proposito,

È una questione importante su cui ci siamo lungamente soffermati in Commissione. Mi riservo poi di riparlarne in sede di illustrazione degli emendamenti. È evidente che l'articolo 11 del disegno di legge al nostro esame, che contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive del cosiddetto pacchetto Telecom, risulta però troppo generica ed a mio giudizio appare evidente la necessità di rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. In tal senso, va l'emendamento 11.202 da noi presentato. Un altro punto rilevante della legge comunitaria riguarda l'articolo 12, che risponde alla continua crescita della domanda di consulenze professionali relative all'*asset protection* con un nuovo strumento, il contratto di fiducia. L'obiettivo è naturalmente quello di limitare il ricorso ai *trust* di diritto estero ed aggiornare l'ordinamento interno adeguandolo ai principi dell'Unione europea. Nella relazione di accompagnamento al provvedimento, ciò si è reso necessario sulla base del fatto che nell'ultimo decennio il mercato italiano ha registrato un costante incremento di richieste di prestazioni legali e più ampiamente professionali inerenti ad operazioni fiduciarie. Negli ultimi anni il *trend* ha comportato in larga misura la ricerca di soluzioni basate sul ricorso al *trust.* La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sul riconoscimento dei *trust* ha dato il "la" al dipanarsi di giurisprudenza, prassi e dottrina italiane sulla materia. La relazione governativa sottolinea però che, nonostante quest'apertura, la Convenzione «non impone affatto all'Italia l'obbligo di riconoscere *trust* interamente localizzati sul nostro territorio. Più semplicemente, l'operatore italiano si è rivolto al *trust* retto dalla legge straniera a causa dell'assenza nel diritto italiano di un istituto equivalente sotto il profilo della completezza, della flessibilità e della coerenza interna delle norme che lo regolano». motivo il legislatore ha cercato di trovare un rimedio nel 2005, con l'introduzione nel codice civile dell'articolo 2645-*ter*, riguardante la trascrizione dei vincoli derivanti da atti di destinazione: una scelta certamente ispirata dalla volontà di arginare il ricorso alla legge straniera da parte di soggetti italiani. Ora, a cinque anni di distanza, per allineare l'ordinamento nazionale ai principi del diritto dell'Unione europea, l'Esecutivo intende implementare un nuovo istituto giuridico, il contratto di fiducia appunto, mutuandolo dal sistema francese. Nel 2007, il legislatore transalpino ha infatti previsto nel proprio diritto la "fiducia", con la finalità di mettere a disposizione degli operatori uno strumento competitivo rispetto ai *trust*, sia dal punto di vista delle operazioni fiduciarie di *asset management*, sia per quanto attiene all'*asset protection* (va ricordato, peraltro, che la Francia non ha ratificato la Convenzione dell'Aja). Con il contratto di fiducia, che sarà introdotto nella disciplina civilistica italiana, un soggetto (fiduciante) trasferisce beni, diritti o denaro ad un altro soggetto

tuttavia che si è in presenza, da un lato, di una regolamentazione normativa e di prassi abbastanza chiara in materia di imposizione sul reddito, mentre dall'altro sussistono invece incertezze in materia di imposizione indiretta (mi riferisco alle imposte d'atto e di successione e donazione), su cui il legislatore deve intervenire per evitare che lo strumento sia destinato ad una ben limitata operatività.

in materia di tassazione immobiliare. Sarà inoltre necessario distinguere tra contratti di fiduciari riconducibili alla fattispecie del *trust* e contratti di fiducia realizzati a scopo di garanzia, spostando il momento impositivo dallo spossessamento al trasferimento del bene al creditore o al terzo e solo laddove tale trasferimento si realizzi per effetto dell'escussione della garanzia. Questi contratti, per loro natura, dovranno dunque costituire uno strumento agile in uso agli operatori economici per consentire aperture di credito garantite. In conclusione, va detto che la legge comunitaria rappresenta sempre e comunque un momento di viva e consapevole partecipazione del Parlamento al processo di integrazione europea, fine di assolvere agli impegni assunti in sede comunitaria nel rispetto delle specificità di ordine giuridico, istituzionale, economico e sociale del contesto nazionale. È quindi da considerare e da vivere non come un adempimento burocratico fatto esclusivamente per non incorrere in pesanti sanzioni, ma come un provvedimento che costituisce uno dei passaggi finora di maggiore importanza

Grazie e benvenuti.

che nel prosieguo potrà facilmente prestarsi a divenire un contenitore*omnibus* di disposizioni eterogenee. È un'ipotesi tutta da scongiurare, perché così si snatura l'obiettivo stesso per cui la legge era stata concepita, quello di adempiere rapidamente agli obblighi comunitari e fare di più, soprattutto sotto il profilo qualitativo della politica europea. In quanto componente dell'8a Commissione permanente, mi limito qui ad evidenziare alcuni aspetti. Il parere che la Commissione ha reso prima ancora che il Governo e il relatore introducessero, nel corso dell'esame della 14a Commissione, è incentrato sulla norma che reca i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento del cosiddetto pacchetto Telecom. Su questo punto voglio concentrare la mia attenzione al fine di riflettere sulla necessità di non ripetere nel provvedimento gli errori già commessi in precedenza. Mi riferisco in particolare all'indeterminatezza nella delega o all'eccesso di estensione della delega, per cui il Governo può in ogni momento modificare la legislazione. In tal senso, l'articolo 11 reca una definizione di principi e di criteri decisamente poco puntuale, aprendo così possibili pregiudizi agli utenti/consumatori in termini di accesso alla cultura e ad Internet, nonché di garanzia di*privacy*. Il recepimento delle direttive n. 136 e n. 140 del 2009, in materia di comunicazioni elettroniche, è di particolare importanza poiché in esse sono contenuti un insieme di principi strategici e fondamentali per il futuro della rete e dell'innovazione del nostro Paese. Il settore delle telecomunicazioni è l'emblema di quel connubio che la dottrina definisce come il difficile matrimonio tra regolazione e concorrenza. L'articolo 11 indebolisce fortemente la portata del principio della concorrenza, nella misura in cui la lettera *n)* del comma 3 prevede che la definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica avvenga nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare e comunitario di settore e - questo è il punto - nel rispetto della specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali. Successivamente, alla lettera *p)*, viene anche disposto che la valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenga conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale. Passando poi alla disposizione che rafforza le prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, soprattutto in termini di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, occorre evidenziare che la portata della norma è eccessivamente di basso profilo, se confrontata con quanto espressamente previsto dal dettato delle direttive che si dovranno recepire. In relazione ai diritti degli utenti, infatti, il nuovo pacchetto di direttive comunitarie opera un richiamo espresso ai principi di trasparenza e completezza delle informazioni sulle condizioni economiche e tecniche dei servizi offerti. In particolare, tali principi, sanciti a livello normativo, sono da intendersi, tra l'altro, in termini di facilità di consultazione, chiarezza, comparabilità, adeguatezza e aggiornamento dei dati relativi ai prezzi e alle tariffe, nonché, più in generale, alle condizioni vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti. Le autorità possono imporre ai gestori di servizi di comunicazione elettronica di fornire, anche in sede di sottoscrizione di contratti con l'utente finale, informazioni su aspetti rilevanti quali, per esempio, le procedure di misurazione e strutturazione del traffico di reti utilizzate per evitare la saturazione e il superamento di limiti di capienza; le ripercussioni in termini di qualità del servizio; le modifiche alle condizioni che limitano l'accesso; l'utilizzo di servizi e applicazioni. Di tutto questo non vi è traccia nel disegno di legge al nostro esame. La tutela della libertà di comunicazione e la trasparenza delle condizioni di offerta dei servizi rappresentano irrinunciabili obiettivi per lo sviluppo di una società dell'informazione, come è quella del terzo millennio. Mi Mi rammarico del fatto che nel corso dell'esame della Commissione il Governo, che ha pure presentato emendamenti recanti interi nuovi articoli, non abbia provveduto ad accogliere rilievi eccepiti dalla 8a Commissione relativamente all'opportunità di adottare misure volte a promuovere investimenti efficienti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, di prevedere l'obbligo per lo Stato di perseguire le cosiddette buone pratiche in termini di innovazione tecnologica, tra l'altro, già sperimentate a livello regionale. regionale. Credo che soprattutto oggi, con le condizioni precarie che affliggono le famiglie italiane, non ci possiamo permettere di perdere l'occasione di quel motore di sviluppo che passa attraverso la comunicazione elettronica. Con senso di responsabilità senza polemiche futili, chiediamo al Governo e alla maggioranza atti concreti in tal senso.

qualità e nella tipicità dei nostri prodotti, che sono riconosciuti a livello mondiale, ma, se verranno contaminati dagli organismi geneticamente modificati, sarà la fine della nostra agricoltura.

ci troviamo ad affrontare l'esame del disegno di legge comunitaria 2010 in un contesto di grave crisi economica del continente europeo e ad un anno dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Tra gli strumenti che abbiamo a disposizione per superare questo passaggio critico e per consentire all'Italia un pronto adeguamento alla normativa comunitaria, vi è, come noto, anche il disegno di legge comunitaria annuale. Quello che abbiamo di fronte, relativo all'anno 2010, si atteggia come un provvedimento che le Camere devono adottare con un ritardo limitato rispetto, appunto, all'anno di riferimento. Al riguardo, ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento provveda, entro un tempo celere, all'adozione del disegno di legge, in maniera che le Camere possano esaminare la legge comunitaria per il 2011. Inoltre, questo provvedimento si caratterizza per avere una struttura ed un contenuto snelli, in quanto è composto da soli 18 articoli nel testo licenziato dalla 14a Commissione, rispetto a quello della legge comunitaria 2009, che - come si ricorderà - conteneva oltre 50 articoli, nella sua versione definitiva, nonché numerose questioni problematiche. La ragione e il merito della natura leggera di questo disegno di legge comunitaria vanno individuati, essenzialmente, nell'atteggiamento assunto dai componenti della Commissione per le politiche dell'Unione europea durante il relativo esame, nonché - occorre riconoscerlo - nella condotta della Presidenza, improntata, d'intesa con tutti i Gruppi parlamentari, ad una disamina rigorosa dei principi che disciplinano la declaratoria di ammissibilità degli emendamenti. Eguale saggezza è stata dimostrata da tutti i componenti della Commissione in occasione dell'unico momento problematico incontrato nel percorso del disegno di legge presso la Commissione, ovvero quando il Governo ha presentato un apposito emendamento volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2009/43/CE concernente il commercio dei prodotti d'arma. In tale frangente, grazie al contributo fondamentale del rappresentante del Governo, sottosegretario Vincenzo Scotti, si è riusciti a disinnescare il delicato problema connesso all'obbligatoria attuazione della direttiva stessa e alla concomitante necessità di non intaccare i principi generali della legge n. 185 del 1990. Credo che la mediazione raggiunta sia in grado di contemperare i diversi interessi in gioco e consentire all'Italia di ottemperare all'adempimento comunitario che ci chiede di adeguarci a tale atto legislativo entro giugno 2011. Cionondimeno, mi preme richiamare l'attenzione sulla circostanza per cui la legge comunitaria 2010 - pur non presentandosi appesantita da una congerie di disposizioni tra di loro disomogenee - contiene una serie di disposizioni che provvedono a recepire direttive comunitarie riguardanti importanti settori dell'economia. Mi riferisco, tra gli altri, alla disciplina sulla fiducia, alle comunicazioni elettroniche, alle guide turistiche e agli OICVM (organismi di investimento collettivo sui valori mobiliari). Desidero, infine, spendere alcune parole sulla legge comunitaria quale strumento ordinamentale ormai consolidato per il periodico adeguamento del diritto italiano a quello comunitario. Come è noto, sono state presentate, soprattutto presso la Camera dei deputati, alcune proposte legislative - tra cui una di origine governativa - miranti a riformare la cosiddetta legge Buttiglione del 2005. A mio avviso, si tratta di iniziative significative in quanto è opportuno, dopo oltre cinque anni, pervenire ad una sorta di "tagliando" della cosiddetta legge ordinamentale, che regge le modalità di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Sotto tale profilo, quindi, occorre guardare con attenzione alla proposta governativa che prevede un *decoupling*, ossia una sorta di sdoppiamento della stessa legge comunitaria in due distinti atti legislativi, uno contenente la sola delega parlamentare e l'altro di mera novazione legislativa. Tale accorgimento potrà risultare utile, comunque, solo nella misura in cui sarà in grado di accelerare i tempi dell'*iter* parlamentare della legge comunitaria e, conseguentemente, di ridurre il numero e la qualità delle infrazioni comunitarie dell'Italia.

non è fuori contesto, anche se forse alcuni potranno ritenere che parlerò d'altro.

in particolare in questo momento o in questo lunghissimo periodo, è vero che essere a posto, essere in ordine conferisce un dato di credibilità in più. più. È difficile richiedere alle istituzioni europee un'attenzione a qualche settore importante del nostro Paese

che la questione di non avere un Ministro degli affari europei con piena competenza, non soltanto per quanto riguarda la trasposizione nel diritto interno ma anche di stimolo dell'altra funzione, quella di dare idee, al di là e non solo del mercato interno (che già sarebbe molto, considerato che l'applicazione del mercato interno è lungi dall'essere completa)

in una visione più federalista, di un bilancio comunitario all'altezza dei tempi. O l'Europa riesce a farlo, oppure credo che anche questa crisi finanziaria, che ha dimostrato la debolezza e i ritardi europei,

Ho proposto un dato di federazione leggera: non credo vi sia alcuna esigenza di avere un bilancio comunitario del 20 per cento del PIL, sul modello degli Stati Uniti d'America,

Penso che il Governo possa e debba riflettere sulla proposta di un'iniziativa da assumere a livello europeo, perché la pura continuazione dello *status quo*

l'indispensabile elemento per avere - se lo si vorrà - un'Europa credibile, se non in politica internazionale in senso lato,

dal progetto di Barcellona all'Unione per il Mediterraneo e ad altri progetti velleitari, quando non fantasiosi, di fatto si è rivelata fallimentare. Non si tratta di guardare con il retrovisore facendo la critica al passato, cosa peraltro molto facile e su cui ci si può sbizzarrire: si tratta però di capire che la sponda Sud del Mediterraneo ha voltato pagina, comunque la si voglia pensare,

difficilmente presentabile, per non fare nomi - ma una politica che sappia accompagnare libertà, diritto e Stato di diritto ad uno sviluppo economico che fa bene non soltanto ai Paesi, ma perfino, stabilmente, alle nostre imprese. Queste sono le due sfide - lo dico ai colleghi e al Governo - di fronte alle quali è inutile scappare, perché comunque ci inseguiranno. cambiare ed essere all'altezza di queste sfide, con tutti i rischi che ciò comporta, forse possiamo avere la speranza di tornare ad assumere un ruolo, almeno nelle aree che ci circondano.

settore veramente cruciale per la politica europea, che è l'agricoltura. Conosciamo - l'ha citato il senatore Vallardi - l'importante legge sulla etichettatura.

tutti poter estendere questa norma ad un numero maggiore di prodotti. Senatrice Pignedoli, il settore agricolo è sicuramente centrale.

La senatrice Licastro Scardino ha illustrato molto bene quali sono le proposte di modifica della legge n. 11 del 2005, che - come già detto - sono assolutamente necessarie.

le regole finanziarie. Ho trovato molto interessante la sua osservazione in merito alla necessità di dare maggiore importanza alla politica euromediterranea.

il partenariato orientale, che ha eclissato l'euromediterraneo, ha succhiato fondi da quella che poteva essere la politica euromediterranea, senza tenere in minimo conto il fatto che ci sono Paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, Malta e la Grecia per i quali il Nord Africa rappresenta l'altra sponda del Mediterraneo: è su questi Paesi che maggiormente dovremmo lavorare.

sia sempre presentata, fin dal momento in cui è nata, con un'attrattività particolare proprio per i suoi valori di libertà e di democrazia: eravamo un passo avanti rispetto a tutti gli altri Paesi. Ricordo anche, però, rispetto a quanto sta avvenendo nei Paesi del Nord Africa, che un po' di circospezione

adottate alcune riforme, è stato permesso a Khomeini di rientrare e, dopo quattro mesi, lo stesso Khomeini ha condannato a morte il presidente che aveva permesso di fare

Concludo dicendo che l'Europa ha un modo per essere forte e per proporsi in questo in questo mondo globalizzato come un punto di riferimento. Però, per fare questo, io credo che debba essere molto ben radicata e molto ben convinta delle sue radici. Faccio un esempio. Ieri, al Consiglio europeo dei Ministri degli affari esteri, per essere del tutto *politically* *correct*, non si è avuto il coraggio di approvare

le violenze avvenute contro le comunità cristiane in Medio Oriente. Qualcuno ha detto che questa risoluzione avrebbe potuto scatenare una una guerra di religione. Non credo che sia così, e credo che, fino a quando l'Europa non avrà il coraggio delle sue radici e delle sue convinzioni, non andremo assolutamente da nessuna parte.

parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, professor Scotti, al quale chiedo anche di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intende accettare.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di un'ora per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul

osservando che il criterio di delega, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, appare potenzialmente lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali. Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 11.0.301, limitatamente al comma. 2, lettera 14.300 e 14.200, limitatamente al comma 2-*bis*, lettera *d)*, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

illustro l'emendamento 1.100, con il quale si intende togliere dall'elenco delle direttive che devono essere attuate la cosiddetta direttiva rimpatri, una direttiva che sta causando seri problemi all'azione di contrasto all'immigrazione irregolare. Alcune procure della Repubblica, dando una interpretazione a nostro avviso non corretta del provvedimento comunitario, hanno dato indicazioni alle polizie giudiziarie di non procedere all'arresto di clandestini recidivi, quelli cioè che sono già stati oggetto di un ordine di allontanamento. Riteniamo opportuno che su questo tema così delicato e importante ci sia un intervento preciso e specifico del Governo, che sta già già valutando attentamente la situazione sopravvenuta. Ripeto, è una situazione particolarmente preoccupante, anche alla luce di quanto sta accadendo nei Paesi vicini a noi (mi riferisco all'Egitto e alla Tunisia). Quindi, dobbiamo fare in modo che l'apparato sanzionatorio in materia di immigrazione irregolare sia un un apparato il più possibile rigido e rigoroso. In caso contrario, rischiamo davvero l'invasione di flussi migratori illegali. motivo, con questo emendamento chiediamo di fare un piccolo passo indietro, per fare poi un grande passo in avanti con un nuovo provvedimento che possa affrontare completamente in maniera coordinata e organica questo tema così delicato. *(Applausi dal

questo emendamento, che è molto importante. Soprattutto, è importante che sia compresa la procedura con la quale si è arrivati al testo. La direttiva non era presente originariamente

a cui una forza di Governo dovrebbe tendere. E una forza di Governo momentaneamente all'opposizione, come la nostra, ha fatto la proposta

questo emendamento è di fatto il frutto del dissociarsi di due membri di un Gruppo parlamentare rispetto alle scelte del Ministro dell'interno.

possano riflettere i due colleghi della Lega Nord che hanno fatto questa scelta.

votati in Commissione nel mese di novembre, prima che si verificassero nel Paese alcuni fatti che sono stati testé illustrati. Detto questo, credo che l'intento del Ministero dell'interno sia quello di andare al più presto ad un provvedimento, anche attraverso un decreto-legge, per recepire la direttiva e armonizzarla nella legislazione italiana. Quindi, per quello che mi riguarda, il parere è favorevole

che potrebbero non ricordare questo passaggio, vorrei segnalare che la distinzione tra gli allegati A e B risiede nel fatto che il procedimento per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari decorsi 40 giorni,

la ragione di questo emendamento 2.2 è molto semplice: esso nasce dalla preoccupazione che con questa disposizione si proponga una delega generica, in bianco, per l'imposizione di sanzioni. Vi è un oggetto non identificato, vi sono principi di carattere generale e la soluzione finisce per non essere conforme alla previsione dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 11 del 2005 che, pur prevedendo la possibilità di delega, presuppone una più precisa delimitazione della materia e dei criteri. Questa delega, così come formulata e reiterata nel tempo, finisce con l'alterare un equilibrio costituzionale, trasferendo la competenza al Governo in materia di legislazione e con l'applicazione di sanzioni penali o amministrative con riferimento a un criterio molto generico, quello dell'offesa a interessi costituzionali, in maniera tale che il Governo legiferi e la funzione di controllo sia attribuita impropriamente al Parlamento. In questo modo si toccano ancora una volta le prerogative costituzionali del Parlamento.

Presidente, l'ordine del giorno G5.100 pone un tema molto serio per il nostro Paese, che riguarda la tutela giurisdizionale dei cittadini italiani davanti alla Corte internazionale di giustizia e altre problematiche. In estrema sintesi, si è verificato nell'anno passato, nel 2010, che a fronte di una iniziativa giudiziaria di un cittadino italiano che aveva ottenuto una condanna dello Stato tedesco per il risarcimento del danno dovuto ad un crimine di guerra (per la precisione, una sentenza della Corte di cassazione greca per le le vittime della strage della Wehrmacht del 1944 in Grecia), il Governo italiano, dopo che questo cittadino aveva pignorato un bene immobile di proprietà dello Stato tedesco in Italia, ha emanato un provvedimento legislativo (un decreto-legge poi convertito in legge, nel disinteresse generale, evidentemente) finalizzato a paralizzare l'efficacia di questa condanna per un crimine di guerra. Si è cioè stabilito che, ove uno Stato estero ricorra avanti alla Corte internazionale per accertare l'immunità giurisdizionale dello Stato estero, il cittadino non può proseguire l'azione esecutiva e il procedimento è sospeso *sine die* fino a quando la questione non viene risolta. Il nostro Paese inoltre (questa è la ragione per la quale questo tema viene introdotto in occasione dell'esame della legge comunitaria), a differenza di tutti gli altri Paesi europei, non attribuisce ai cittadini italiani la tutela giurisdizionale nei procedimenti davanti alle Corti internazionali finalizzati ad accertare l'immunità giurisdizionale degli Stati esteri. I cittadini italiani non possono stare in giudizio perché nel giudizio tra due Stati la persona fisica non può stare in giudizio a mezzo di un proprio difensore e non può avvalersi della tutela legale del proprio Stato (in questo caso dello Stato italiano), a differenza di ciò che avviene - ripeto - in tutti gli Stati europei. Ciò significa che i numerosissimi procedimenti giurisdizionali per crimini di guerra che sono pendenti sono destinati ad una navigazione incerta e ad un esito che non si sa quale sarà. I cittadini che otterranno la condanna, con ogni probabilità non avranno soddisfazione dei loro crediti fino a quando la questione non sarà risolta. molto seria, con un ordine del giorno si chiede al Governo di riesaminare questo tema e di verificare la possibilità di superare questa norma che ha paralizzato le iniziative esecutive nei confronti degli Stati esteri nelle more della definizione dei giudizi davanti alla Corte di giustizia e soprattutto di attribuire ai cittadini italiani la tutela che loro spetta in giudizi aventi questo oggetto. Chiedo al Governo e alla relatrice particolare attenzione su questo ordine del giorno. Presidente, il parere è contrario, in quanto l'ordine del giorno vanificherebbe lo scopo di una legge,

quindi, quanto mai inopportuno un intervento nelle more dell'ormai prossima decisione della Corte sul ricorso della Germania contro l'Italia. Questa è la ragione molto semplice

si accoglie l'ordine del giorno perché vanificherebbe la legge. La legge ha determinato una situazione a mio modo di vedere insostenibile e l'ordine del giorno in esame è finalizzato a sollecitare il Governo a superarla. Inoltre, la definizione del procedimento che il sottosegretario Scotti assume essere imminente (e mi auguro che sia veramente così, ma bisognerà verificarlo) non risolve il problema più generale, che è quello della tutela dei cittadini italiani davanti alla Corte di giustizia. È evidente che tutti gli Stati stranieri saranno abilitati a promuovere, anche pretestuosamente, un giudizio davanti alla Corte di giustizia per paralizzare l'efficacia esecutiva delle sentenze

parere contrario per le stesse ragioni espresse dalla relatrice. arriviamo ad un paradosso. Questo emendamento è volto alla soppressione della modificazione del codice del consumo introdotta dalla lettera *c)* dell'articolo

è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento» e che l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale reca l'ordinamento transitorio di Roma capitale, la norma in questione prevede la sottrazione del territorio di Roma capitale dal NUTS 3 comprendente tutta la provincia di Roma, elevandola al rango del NUTS 2, oggi riconosciuto alle Regioni, così da renderla un'area da ricomprendere nell'obiettivo 1. Si ritiene che il Governo debba procedere ad un'operazione di questo tipo nell'alveo della successiva decretazione prevista per l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

siamo favorevoli, essendo una forza che aspira a governare, a che Roma come area metropolitana abbia la possibilità di accedere, come accade per Berlino, Parigi e Londra, ai fondi come se si trattasse

quello vero: trasformare le aree metropolitane in Province metropolitane. Quindi, la nostra è una dizione quasi terminologica, ma che dà sostanza a questo fatto. altrimenti esprimo parere contrario, in quanto ricordo che nella legge n. 42 del 2009 il territorio di Roma capitale corrisponde a quello del Comune di Roma, che costituisce appunto la sua area metropolitana.

approvò un ordine del giorno che mirava a sanare un paradosso che sembrava quasi impossibile potesse accadere. L'integrazione europea è passata per gradi, attraverso la libera circolazione delle merci, successivamente

nei vari Paesi membri si rilascino dei brevetti o abilitazioni sulla base di criteri indubbiamente diversi. Un maestro di sci abilitato all'estero può comunque, per l'accordo economico esistente, insegnare la materia anche in Italia.

Colleghi, per cortesia, evitiamo

Presidente, illustro gli emendamenti a mia prima firma, che sono sostanzialmente riassumibili

di evitare che, attraverso il recepimento di direttive comunitarie - non è accaduto solo questa volta - si stravolgano alcune regole ormai acquisite per quanto riguarda: la neutralità della rete e la sua apertura; la non discriminazione dei soggetti che afferiscono alla stessa rete; il ruolo delle autorità indipendenti;

utili a rimettere in ordine gli addendi, nel senso che la normativa comunitaria non può essere stravolta nei fatti sulla materia della comunicazione,

il rappresentante del Governo a riflettere bene su questi emendamenti, che non sono altro che l'applicazione più fedele della normativa comunitaria, così come avviene anche in altri Paesi.

11.202, a firma Germontani, Saia e Pedica, riguarda il rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'inserimento della lettera *0a)* è

La necessità di colmare tale lacuna deriva dalla circostanza che detto principio è invece espressamente previsto dalla direttiva Quest'ultima sottolinea proprio l'esigenza che nelle legislazioni nazionali sia prevista una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione, responsabile *ex ante* del mercato e della risoluzione di controversie tra imprese, sia al riparo nell'esercizio delle sue funzioni da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità dì giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere. È quindi necessario che il principio di indipendenza sia garantito anche con riferimento alla nomina dei membri dell'organo collegiale, anche in considerazione di quanto previsto da altre autorità di regolamentazione in ordine alla nomina dei propri Quindi, l'intervento che proponiamo elimina lo specifico riferimento al mercato, non essendo la locuzione «accesso al mercato» prevista da alcuna disposizione di cui alla direttiva

che le vengono esplicitamente attribuite dalla direttiva 2002/20/CE, e questo attraverso l'intervento emendativo al comma 3, lettera *q)*.

nell'informazione, per garantire accesso paritario e non discriminatorio e per far sì che Sky, La7 e tutte le altre più piccole emittenti televisive (piccole ma libere) ma libere) abbiano uguali diritti e non subiscano la tirannia, né del conflitto di interessi Mediaset, né della politicizzazione delle telecomunicazioni RAI. L'Autorità è stata portata alle cronache qualche mese fa, come sapranno tutti i colleghi, a causa di pressioni esercitate dal Presidente del Consiglio sul consigliere Innocenzi, al fine di chiudere alcuni programmi scomodi per l'Esecutivo, come «Annozero» e «Parla con me», e di zittire le voci più critiche, come quella del presidente Di Pietro. Per questo, condivido totalmente l'intento e le finalità dell'emendamento proposto dalla collega Germontani e chiedo ai colleghi di votare a favore, garantendo una maggiore indipendenza dell'Autorità, in quanto un'informazione pubblica, equa ed imparziale è prezioso fondamento del nostro tessuto democratico.

Sen.

**Il Senato non approva.**

relatrice. Questi emendamenti, che vengono tranquillamente - e un po' mestamente - respinti, sono emendamenti utili a evitare un ginepraio interpretativo della normativa italiana sulle comunicazioni. Vi prego solo, per sincerità, di dare un'occhiata a questi testi, che non sono di parte: sono testi che provano a rendere compatibile la normativa italiana con quella comunitaria. Quindi, sarebbe interessante che la *routine* prendesse anche atto, ogni tanto, dei contenuti.

Presidente, per quanto attiene all'emendamento 11.212, sarei davvero incuriosito da ogni punto di vista

a semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese, cosa che chiunque abbia messo il naso in questo settore della comunicazione sa che è un problema. È innocuo questo emendamento! Mi chiedo perché ci

chiede al Governo e alla maggioranza di mantenere quelli che furono i soliti impegni presi in campagna elettorale - non ricordo quale fosse l'anno, ma insomma, tutte le volte ce n'è una! prima di passare alla persecuzione dei rom e degli immigrati, c'era infatti la promozione dell'impresa, di Internet e dell'inglese. Il risultato è che si dà parere favorevole ad un ordine del giorno in cui si prevede che - per carità, senza toccare le casse dello Stato - bisogna stare attenti ai disagi derivanti addirittura dall'inquinamento elettromagnetico per i Comuni che installano le reti, salvo poi non promuovere la banda larga e dimenticarsi

di comunicazioni elettroniche arriva addirittura ad introdurre il principio del diritto all'accesso alla rete per i cittadini dell'Unione europea, stabilendo la cosiddetta neutralità della stessa come principio necessario non solo a garantire i diritti civili degli utenti della rete compreso, appunto, quello all'accesso - ma anche le garanzie di un libero sviluppo del mercato delle telecomunicazioni e, in generale, dell'economia dell'informazione. Vi è poi tutta la questione della redistribuzione di ciò che è avvenuto con il passaggio dall'analogico al digitale, per cui si cerca in qualche modo di aprire quanto più possibile il mercato a frequenze che sono

promozione sia dell'impresa che di Internet, ed essendo Internet qualcosa, già nel nome, non necessariamente autarchico, anche dell'inglese. Per esempio si chiedeva, e si continua a chiedere, con la speranza che ci si ripensi: di implementare la rete di banda larga e ultralarga, con l'obiettivo di raggiungere la totalità dei cittadini entro il 2015; di procedere alla messa in gara di parte delle frequenze che si liberano nel passaggio dalla televisione analogica a quella digitale; di implementare il diritto di accesso contenuto nella direttiva, garantendo concretamente l'accesso alla banda larga a tutti cittadini italiani come diritto fondamentale, dando a tutti gli operatori del mercato la possibilità di contribuire al soddisfacimento di tale diritto; di garantire che eventuali restringimenti di accesso siano vincolati a procedure eque e imparziali, garantendo in ogni caso il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo; di garantire un accesso non esclusivo allo spettro radio; di difendere la neutralità della rete, innanzitutto garantendo adeguata trasparenza anche rispetto a pratiche di *traffic shaping* volte a privilegiare o a filtrare alcune applicazioni e contenuti (quindi anche questioni relative alla libera concorrenza); di includere - richiesta molto importante visto e considerato che esistono in Italia anche persone diversamente abili e la popolazione è una tra le più vecchie al mondo - nelle apparecchiature terminali cui garantire l'accesso, in particolare a disabili, anziani e soggetti con esigenze sociali particolari, anche gli strumenti necessari ad esercitare la cosiddetta democrazia elettronica e, infine, di rafforzare le prescrizioni anche in ordine ai tempi e alle modalità di cancellazione dei dati personali (anche questa è un'ulteriore decisione presa dall'Unione europea). Ora, è stato espresso un parere, anche perché, ritengo sicuramente per un puro caso (il caso alle volte fa bene le cose; questa volta no), il nostro ordine del giorno non era all'interno del fascicolo, e quindi non c'è stato tempo per poterlo studiare. rivedere in senso positivo il parere espresso su questo ordine del giorno e dare anche un segnale (visto e considerato che nel prossimo pacchetto sicurezza si dovrebbe andare ad abolire il cosiddetto decreto Pisanu) per favorire o per porre meno ostacoli possibili alla promozione di Internet,

Sappiamo che i dati relativi al voto restano agli atti. Bene, ci sono voti che variano di quattro o cinque unità a seconda dell'emendamento, perché ci si accorge magicamente che c'è o non c'è il detentore della tessera.

mi interessa sottolineare soprattutto che il diritto comunitario mi sembra oggettivamente diventato una fonte di diritto primario, che forse necessiterebbe da parte di tutti un'attenzione maggiore e soprattutto di riforme radicali dell'ordinamento italiano, perché si possa garantire un recepimento di qualità tempestivo ed efficace, cosa che, come abbiamo visto anche oggi, non Siamo ancora, io penso, in presenza di intralci oggettivi che negano aprioristicamente la possibilità che ciò possa avvenire. Uno dei maggiori intralci è sicuramente costituito da un'assenza politica di questo Governo nella dimensione europea, e soprattutto a partire dalle questioni che abbiamo di fronte a noi. Mi riferisco, in particolare, alla questione euromediterranea. Siamo di fronte a un Governo immobile che sta procurando enormi danni al Paese, ma non c'è solo questo. C'è anche, a mio modo di vedere, un intralcio dovuto all'interpretazione che viene puntualmente data dalla Commissione bilancio dell'articolo 81 della Costituzione, e cioè che il recepimento non debba prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo stato attuale, la relazione tecnica di accompagnamento della legge comunitaria conferma la consueta modalità di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2, comma 1, che, nei casi di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento, prevede che non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti

vorrei rammentare a tutti noi che la nuova legge di contabilità, all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, stabilisce che, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione di questi ultimi, previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di copertura. Ricordo, inoltre, che la copertura di eventuali oneri a valere sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, appare analoga a quella presente nelle precedenti leggi comunitarie a decorrere dall'anno 2007.

da noi presentati prima in Commissione e poi in Aula, prevedono disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di Paesi terzi trattenuti di poter entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari, nonché ad assicurare la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti. Come possiamo vedere, si tratta di diritti che si sostanziano in strumenti già esistenti per i cittadini italiani che, quindi, vanno semplicemente estesi ai cittadini dei Paesi terzi, con un costo esiguo e, peraltro, coperto anche da fondi europei. Risulta perciò, sempre a mio modestissimo modo di vedere, privo di fondamento il parere della Commissione bilancio per il quale questi emendamenti debbono essere aprioristicamente dichiarati improcedibili ai sensi dell'articolo 81 In questo modo, cari colleghi, si crea una contraddizione: da una parte riconosciamo una base di diritti minimi ai cittadini di Paesi terzi, così come previsto dalla direttiva che andiamo a recepire; dall'altra, e contemporaneamente, li neghiamo nella pratica. Questo sistema, che apparentemente è coerente con la difesa del controllo dei conti, in effetti si rivela un *boomerang* perché ci espone viceversa a sostenere non solo i costi dell'infrazione, ma anche quelli sociali che derivano da questo genere di recepimento. In questo, ascrivo l'atteggiamento, anche oggi, dei colleghi della maggioranza e del Governo nei confronti della direttiva sui rimpatri. Non si tratta, quindi, di un'interpretazione capziosa della sottoscritta, ma di una questione rilevante, e proprio per questo avrebbe bisogno di tutta l'attenzione. È anche lo stesso Servizio del bilancio del Senato che ha iniziato a porsi le stesse perplessità. Voglio perciò sottolineare che l'applicazione automatica dell'articolo 81 della Costituzione ad uno strumento di mero recepimento di diritto sovranazionale, che si attua solo attraverso la delega al Governo, diventa un ostacolo alla libera espressione della volontà del Parlamento, oltre che un esercizio di controllo puramente formale, non potendo il Parlamento esprimersi sui decreti legislativi di attuazione, attualmente - per effetto delle deleghe - nelle competenze esclusive del Governo. una lettura, quella dell'articolo 81, che cozza anche con la legge di contabilità, spingendo verso il non recepimento, o il recepimento parziale, della normativa europea, come state facendo in tutti questi anni di Governo

che stia proprio qui la questione di fondo per cui c'è effettivamente la necessità di voltare al più presto pagina, nel nostro Paese. Vale la pena, in questo senso, ricordare che anche il diritto, ma soprattutto la logica, vorrebbe che, per applicare una direttiva, si mettessero in atto tutti gli strumenti necessari a far rispettare il diritto europeo,

finanziaria. Questo è un meccanismo burocratico e barocco, finalizzato solo ad un recepimento formale, che non regge più ai tempi e che inesorabilmente emargina sempre più l'Italia, anziché favorire un processo di civile e moderna armonizzazione

Penso che la nostra appartenenza all'Unione e tutto ciò che ne discende sul terreno dell'applicazione del diritto debba essere trasparente, coinvolgente e soprattutto non debba essere di parte, per corrispondere adeguatamente all'interesse generale.

rispondano ad una mia interrogazione, sottoscritta anche dal capogruppo della Commissione attività produttive Marco Filippi e dal collega Francesco Sanna, relativamente alla situazione che si è determinata nella compagnia aerea Meridiana Fly. Dal 2 marzo, giorno di presentazione della mia interrogazione, ad oggi le cose sono fortemente peggiorate. È proprio di qualche giorno fa la notizia fornita dagli amministratori della compagnia riguardo alla volontà di quest'ultima di attuare un piano industriale a seguito del quale si dovrebbe procedere al licenziamento di 600 oppure di 800 persone: tale numero incide per più della metà rispetto alle persone attualmente occupate in quella compagnia. Trattandosi di un'azienda di grande prestigio, che assolve ad una funzione di straordinaria importanza, a beneficio, in particolare, della Regione Sardegna, dell'isola della Sardegna,

la prego, signora Presidente, di intervenire con la sua ben nota autorevolezza presso il Presidente del Consiglio e il Ministro a cui ho accennato affinché il Governo ancora in carica voglia prestare attenzione a questo problema così grave. È inaudito che in presenza di una possibile chiusura di una compagnia aerea tutta italiana (non parlo ovviamente dell'Alitalia, ma di Meridiana, che - ripeto - è tutta italiana) il Governo non abbia ritenuto di dover muovere un dito. In questi ultimi giorni dell'impero, fino a quando questo impero ci sarà, è indispensabile, signora Presidente, che chi ha ancora una carica la eserciti, a tutela della Sardegna, della compagnia e degli stessi lavoratori che concretamente rischiano,

praticamente un anno fa - quando indirizzavo, insieme ad altri parlamentari piemontesi, un'interrogazione al ministro Gelmini

un'interrogazione profetica, legata allora ad una mera valutazione di un'inaugurazione, e ora, invece, materia di discussione delle forze politiche cittadine. Ci auguriamo che, a un anno di distanza, il ministro Gelmini, alla soglia della definizione dei nuovi statuti, possa dar conto di questa particolarità tutta sabauda.